la certezza della mobilità nel Paese per gli italiani e per i tanti stranieri che hanno scelto il nostro Paese per le vacanze: ritardi, cancellazioni, bus sostitutivi; aumento dei prezzi alla ricerca drammatica di soluzioni alternative ai trasporti; ritardi di oltre il 20 per cento per i treni solamente nel mese di luglio e ritardi aerei di oltre il 64 per cento rispetto all'anno precedente. Insomma, il Paese è totalmente disconnesso. Purtroppo siamo davanti a un disastro

a recuperare, è grande il caos che ci attende nei prossimi giorni per la modifica della circolazione dei treni a lunga percorrenza. Cito alcuni esempi. La linea AV Milano-Bologna, dal 12 al 18 agosto, cioè nel cuore delle vacanze estive, sarà interrotta

Firenze-Roma, dal 12 al 23 agosto, sarà interrotta in una tratta importante, quella tra Chiusi e Orvieto. Anche in questo caso ci saranno aumenti dei tempi di percorrenza per oltre ottanta minuti. L'Alta Velocità Milano-Venezia: si prevede un'interruzione totale nella tratta Verona-Vicenza fino al 20 agosto. la linea Bologna-Prato, è prevista un'interruzione continuativa di linea fino all'8 settembre. I treni saranno cancellati e sostituiti con bus. In merito ai valichi: sulle linee Milano-Domodossola e Domodossola-Iselle saranno cancellati tutti i collegamenti tra Domodossola e Milano.

disastro, a un'Italia disconnessa, a un'Italia che non riesce in questo momento a connettere le sue città principali, e non riesce neanche a far funzionare i treni regionali. In tutto questo, ci chiediamo - è questo il motivo del mio intervento - dove sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Non lo abbiamo visto in quest'Aula la scorsa settimana, quando lavoravano per convertire il decreto-legge a lui tanto caro, chiamato salva casa, che noi abbiamo ribattezzato salva abusi. Allora non si è degnato di venire in quest'Aula. Oggi, però, il suo silenzio è ancora però, via *social* le sue opinioni sui risultati alle Olimpiadi. Probabilmente, agli italiani serve sapere in che modo si interverrà subito da parte del Governo.

perché i disagi nei trasporti riguardano tutto il Paese. Se dovessimo guardare alle Regioni *top five* come bollino rosso dei trasporti, abbiamo la Calabria, la Toscana, la Campania, il Lazio e il Veneto. In sostanza, hanno unito l'Italia nell'ambito

ferroviario, il Gruppo Partito Democratico chiede che il ministro Salvini venga in Aula a dirci se è capace di dare una risposta al Paese sulle inefficienze che stanno registrando gli italiani e i tanti stranieri presenti nel nostro Paese. *(Applausi)*.

la ringrazio di avere chiarito che la richiesta di utilizzare il mese di agosto per un'informativa immediata del ministro Salvini su quello che sta accadendo nel Paese è stata avanzata

signor Presidente, che noi non possiamo permetterci di interrompere i lavori per la pausa estiva di quest'Aula senza avere dato una risposta seria agli italiani ai turisti che vengono in questo Paese e si trovano con i trasporti al collasso. Peraltro, io sarei anche per dare una risposta rispetto al 15 per cento di spesa che il Ministero delle infrastrutture ha fatto sul PNRR, che è una vera e propria vergogna, perché

recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

rappresentante del Governo, con questo provvedimento ci occupiamo di tutta una serie di opere e investimenti strategici per il Paese, fondamentali per il suo progresso, la sua competitività e la sua crescita economica, che da troppo tempo attendono di essere portati a termine. Il decreto è suddiviso in quattro Capi recanti disposizioni in materia di infrastrutture di interesse strategico, investimenti di interesse strategico, efficienza del procedimento penale e sport. L'articolo 1 reca disposizioni in materia di concessionarie autostradali in particolare, prevede che le concessionarie, per le quali la scadenza del periodo regolatorio quinquennale intervenga nel corso dell'anno 2024, siano tenute a presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari entro il 31 luglio 2024. Poi si modifica la disciplina dell'individuazione del corrispettivo dovuto da ANAS per l'acquisto dei progetti relativi all'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, stabilendo che tale corrispettivo deve essere determinato sulla base di una valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio delle certificazioni di bilancio. Poi si prevedono disposizioni relative alla A22 Brennero-Modena. L'articolo 2, invece, apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 35 del 2023 in materia di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Anche qui, ancora una volta, si interviene con previsioni accelerate dell'*iter*. In primo luogo, infatti, si elimina il termine del 31 luglio 2024 per l'approvazione del progetto esecutivo, prevedendo che l'approvazione invece possa avvenire anche per fasi costruttive. Riteniamo che la possibilità di approvare il progetto esecutivo del Ponte per fasi costruttive progressive - come avviene poi, tra l'altro, per analoghe opere complesse - sia la decisione più idonea per rispettare i tempi di realizzazione, anche in considerazione del gran lavoro che si sta facendo per l'adeguamento del progetto ai nuovi *standard* ambientali e di sicurezza. Si interviene poi anche sotto altri aspetti, e cioè si chiariscono le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione. Si esplicita che il costo dell'opera deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Si chiariscono alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi, e cioè si prevede che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale sia sottoposta ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Poi si specifica ancora che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiano. Si introducono, inoltre, una serie di norme speciali per le procedure espropriative che - da un lato - tutelano il diritto all'abitazione, ma - dall'altro - garantiscono la più celere realizzazione dell'opera, incentivando l'utilizzo degli atti di gestione volontaria anziché delle espropriazioni forzate. C'è un cambio di paradigma che consente a chi vive nelle aree su cui dovrà sorgere il Ponte di non dover subire senza un'effettiva e sufficiente compensazione, e per gli espropri, cosiddetti bonari, per i quali la legge fissa una maggiorazione del 10 per cento, vengono destinati 40 milioni di euro. L'articolo 3 prevede l'adozione di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari per efficientare la loro attività e poi viene istituito, presso il MIT, l'osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali. L'articolo 4 dispone tutta una serie di attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia. L'articolo 5, invece, prevede una serie di interventi volti a sbloccare opere di interesse strategico il finanziamento di interventi che, per svariate ragioni e motivi - prima di tutto per l'aumento dei prezzi delle materie prime e il caro energia, ma anche per altri problemi sopraggiunti - rischiano di non essere completati. di infrastrutture disseminate lungo tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud, che interessano quindi un po' tutta la popolazione e rendono perciò questo nuovo insieme di norme ancora più importante, in quanto va a toccare e a rispondere ai bisogni e agli interessi di tutti gli italiani. L'articolo 6 poi prevede che Cassa depositi e prestiti, previa autorizzazione del MIT, possa erogare entro dicembre 2028 le somme residue relative ai mutui concessi per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali o per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa. L'articolo 8 istituisce presso il MASE il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ e la segreteria tecnica. Nel Capo II, invece, in materia di investimenti di interesse strategico, l'articolo 10 reca misure urgenti per il sostegno della presenza delle imprese italiane nel Continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, si prevede la disponibilità del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, che possono essere utilizzati nel limite di 200 milioni, e per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che sono presenti stabilmente, esportano o si si approvvigionano nel Continente africano o sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenere le spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali ecologici nonché produttivi o commerciali. Si autorizza Cassa depositi e prestiti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti a valere sulla gestione separata, al fine di sostenere iniziative e progetti nell'ambito del Piano Mattei. Nel Capo III si trova poi il solo articolo 11, che reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in Cassazione, finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso. Nell'ambito poi del Capo IV, l'articolo 12 proroga dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale sono eliminate le limitazioni alla libertà contrattuale degli atleti per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023. L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore del

Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, eccoci con l'ennesimo decreto d'urgenza e l'ennesima pregiudiziale di costituzionalità. Se il Governo spera di prenderci per stanchezza, si sbaglia: noi non molliamo mai e il MoVimento 5 Stelle continua, giorno dopo giorno, a denunciare in quest'Aula, per suo tramite, Presidente, agli italiani quel che di vergognoso sta accadendo in Parlamento. Noi non siamo ricattabili, noi no davvero. Noi abbiamo le mani libere e le useremo per difendere la legalità e il rispetto delle regole nell'interesse dei cittadini. Un decreto-legge dovrebbe essere un modo per legiferare, utilizzabile solo in presenza di casi di straordinaria necessità ed urgenza. Invece, per questo Governo esso assurge a metodo di lavoro; un Governo, quello meloniano, che negli atti e nei fatti svilisce il ruolo del Parlamento azzittendolo. Intendo di tutto il Parlamento, maggioranza compresa. L'assioma è il seguente: o si fa come dice il Governo o il Governo cade e porta con sé la maggioranza parlamentare; insomma, prove tecniche di premierato. Ogni forza di maggioranza ha peraltro le proprie priorità, e la pretesa di soddisfarle tutte contemporaneamente porta a un risultato disastroso, privo di un disegno organico, e al susseguirsi della decretazione d'urgenza - ad oggi siamo a settanta decreti

apposizioni di fiducia, con una media di circa tre fiducie al mese; ventuno disegni di legge sono stati approvati con la fiducia di entrambe le Camere, battendo ogni *record* dei Governi che lo hanno preceduto e che hanno governato anche in tempi di pandemia, quando l'emergenza sanitaria globale era, per antonomasia, una condizione di emergenza. Un Governo e una maggioranza prepotenti e supponenti, che paiono animati più da spirito di rivalsa che dal fine di perseguire gli interessi del Paese. Assistiamo a una frenetica corsa contro il tempo per smontare l'impalcatura normativa di chi li ha preceduti, con una produzione normativa abnorme che privilegia la quantità alla qualità, senza valutazioni oggettive ponderate anche dal dialogo parlamentare, che ormai sistematicamente viene aggirato dai decreti-legge e dall'apposizione della fiducia. Gli stessi presidenti Fontana e Centinaio hanno di recente ammesso pubblicamente che occorre ridimensionare il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il ritmo attuale è tra l'altro insostenibile anche per gli uffici tecnici, legislativi e Commissione, costretti a lavorare senza i tempi tecnici per farlo con calma e oculatezza, come la fase legislativa meriterebbe. Questo Governo ricorre al decreto-legge anche quando - come nel caso del decreto in esame - la straordinaria necessità e l'urgenza non siano ravvisabili e motivabili. Infatti, se andiamo a ricercare nel decreto le motivazioni a sostegno dell'adozione di questo *iter* legislativo, che dovrebbe essere l'eccezione, troviamo il vuoto cosmico. Di norma, le motivazioni non si forniscono in due casi: quando non esistono o quando è preferibile non svelarle; nell'uno e nell'altro caso si tratta di un *vulnus* preoccupante, oltre che incostituzionale. Nel preambolo del decreto non vi è traccia di approfondimento e di argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza, come viceversa prescritto dall'articolo 77 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 76, che ammette la possibilità di delega della funzione legislativa al Governo solo con le dovute cautele, in ossequio al principio della divisione dei poteri, che attribuisce la funzione legislativa al Parlamento. Fondamentalmente le motivazioni del preambolo sono tautologiche, cioè alla domanda: perché il Governo ha deciso di intervenire con decretazione di urgenza? La risposta è la seguente: perché sono urgenti. Il Governo risponde al Parlamento come se rispondesse a un bambino troppo curioso. Domanda: perché? Risposta: perché sì. sì. Onorevoli colleghi, qui siamo in Parlamento, qui l'interlocutore sono i rappresentanti del popolo e, indirettamente, il popolo stesso. Può un Governo serio e responsabile argomentare con un «perché sì»? Il decreto-legge è uno strumento eccezionale e la mancanza del presupposto dell'urgenza configura, da un lato, un vizio di legittimità costituzionale del decreto e, dall'altro, un vizio *in procedendo* della legge di conversione. I limiti che la Costituzione pone al ricorso alla decretazione d'urgenza trovano fondamento nel rispetto del principio della divisione dei poteri: quello legislativo al Parlamento e al Governo quello esecutivo. Questi limiti valgono anche come deterrente per evitare «un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto»: sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2024. A nulla paiono però valere i richiami Con questo Governo assistiamo a un disorganico delirio normativo a suon di decreti *omnibus* come quello in esame, in fase di conversione, che reca interventi che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie molto diverse tra loro. Appare dunque evidente che si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza di dubbia legittimità, che ha la pretesa di coniugare in un unico contesto normativo profili di necessità ed urgenza riferiti a materie che non presentano attinenza e coerenza interna e, dunque, carenti altresì del requisito di omogeneità materiale e teleologica, come richiesto dall'articolo 77 della Costituzione. Insomma, è un decreto pastrocchio in cui l'unico *fil rouge* tra le diverse materie è quello di non avere il carattere dell'urgenza; un decreto da stralciare per riprendere invece il percorso legislativo ordinario. L'articolo 8, in tema di Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO₂, stabilisce che parte delle risorse dei proventi delle aste delle quote di CO2, di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, per la quota che verrà assegnata al Ministero dell'ambiente, sarà destinata per la copertura dei costi per i compensi dei membri del Comitato e della segreteria. Purtroppo, il comma 3 dell'articolo 23 stabilisce che i proventi delle aste delle quote di CO2 sono versati alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati su appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante dagli obblighi europei, ai sensi e agli effetti della direttiva 2003/87, ovvero transizione ecologica. Qua, invece, si destinano le risorse a spese correnti per gli stipendi dei membri del Comitato piuttosto che a spese di investimento utili. Parliamo dell'articolo 2, quindi del Ponte sullo Stretto: qual è la straordinaria urgenza per il Paese di investire decine di miliardi nel progetto del Ponte, caratterizzato da un *iter* normativo, solo in ragione della sua durata, di oltre cinquant'anni? Ciò esclude a priori l'ipotesi che ci troviamo di fronte a un intervento infrastrutturale caratterizzato dal connotato dell'urgenza e aggiungerei da quello della costituzionalità. nell'urgenza di portare avanti il progetto, il Governo ha riavviato l'*iter* approvativo interrotto da oltre dieci anni per pervenire, mediante procedimento accelerato e semplificato, all'approvazione del progetto definitivo e stabilendo la sostituzione del progetto esecutivo con un meccanismo di approvazione per stralci funzionali, che consente la realizzazione dell'opera per fasi costruttive e progressive, eliminando la scadenza del 31 luglio, originariamente prevista per l'approvazione del progetto definitivo e rinviando la verifica delle criticità alla fase esecutiva. Come possiamo approvare un progetto senza il progetto definitivo? Lo stesso progettista chiede verifiche preventive per avere la certezza della tenuta dell'opera. La VIA non è stata conclusa; l'Unione europea non ha ancora autorizzato il cofinanziamento per la parte ferroviaria, in quanto non ha certezze sulla tenuta dell'opera e non è considerato l'impatto ambientale dell'opera, in particolare sulla fauna e sul sistema aviario. Vi è di più: quest'opera, oltre a non essere necessaria e urgente, è altresì dannosa. È noto che nello Stretto sia presente una delle più alte concentrazioni di biodiversità al mondo e sussistono gravissime criticità ambientali per l'impatto che l'opera produrrebbe sul delicato insieme di ecosistemi presenti nell'area, con una palese violazione dell'articolo 9 della Costituzione che tutela ambiente, biodiversità, ed ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; vieppiù se letto nel combinato disposto con l'articolo 41, che sancisce che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto all'utilità sociale e in modo da arrecare danno alla salute e all'ambiente. Poi mi chiedo: se si pretende davvero di essere credibili, parlando di urgenza e priorità attuale a proposito della costruzione quando sappiamo che ormai da diverse settimane in Sicilia, come in Calabria e in gran parte del Sud Italia, non c'è acqua per irrigare i campi coltivati, non c'è acqua per dissetare bestiame, non arriva acqua ai rubinetti delle case una parte d'Italia soffre la sete nel 2024, il Governo cosa risponde? È urgente costruire un ponte. Ma se mancano i collegamenti interni, se i treni vanno ancora con il comignolo, il Governo cosa risponde? Facciamo subito un bel ponte e lo decretiamo con urgenza. Spiegateci perché? "Perché sì".

Le risorse delle nostre casse pubbliche sono limitate - lo sappiamo - e devono essere gestite con oculatezza dal buon amministratore pubblico. Per garantire un servizio idrico efficiente occorre pianificare e programmare gli interventi utili con anticipo; occorre investire denaro ora cominciare ora per vedere i risultati tra qualche anno; investire in questo e non buttare in altro risorse. Abbiamo un Nord Italia sommerso da alluvioni e inondazioni e un Sud arso dalla siccità e senza acqua. Le infrastrutture idriche e la prevenzione del dissesto idrogeologico sono la priorità, e non certo un ponte di cui nessuno percepisce la necessità e urgenza,

presentare una questione pregiudiziale sul provvedimento, per una serie di ragioni. Prima di tutto siamo di fronte all'ennesimo decreto-legge che viola sostanzialmente quanto stabilisce la la Costituzione, che viola continuamente il richiamo del Presidente della Repubblica, che viola anche i suggerimenti dati dalla Corte costituzionale. In sostanza, ormai la decretazione d'urgenza avviene su tutto. Vorrei sottolineare, oltre alla messa in discussione del ruolo parlamentare - cosa che denunciamo tutte le volte che c'è una fiducia e c'è un decreto, e purtroppo ogni giorno c'è un decreto, se non due

tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, personale dell'Autorità per la Laguna di Venezia; finanziamento alla fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli; misure in materia di trasporto pubblico locale; bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani; cattura e stoccaggio geologico dell'anidride carbonica; Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico-tecnologico di Genova Erzelli; misure a favore delle imprese italiane all'estero; modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport. Ma secondo voi, oggettivamente, ha un senso questo modo di fare?

per l'interesse strategico di aziende che sono in Africa, che lavorano e operano nel Continente africano? Forse non sarebbe il caso di fare una discussione su questo, visto che parliamo di *made in Italy* e di aiuto a casa loro?

sul decreto-legge che stiamo per convertire, possa essere utile richiamare una recentissima sentenza della Corte costituzionale pubblicata circa dieci giorni fa, che, come probabilmente i colleghi ben sanno, ha dichiarato incostituzionale parte del decreto-legge n. 51 del 2023. In particolare, ha dichiarato incostituzionale la disposizione che prevedeva la cessazione della carica di sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avessero compiuto il settantesimo anno di età. Ha dichiarato incostituzionale questa disposizione per violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Nell'ampia

innanzitutto che, come sappiamo anche noi, l'adozione del decreto-legge è prevista come ipotesi eccezionale ed è subordinata al rispetto di condizioni precise, coerenti con la natura parlamentare della forma di Governo di Governo e con la natura e la funzione che la nostra Costituzione attribuisce al Parlamento, quale unico organo direttamente espressivo della sovranità popolare. Questi limiti, scolpiti nell'articolo 77 della Costituzione, consistono

È cioè condizione di validità del decreto-legge che sussista un caso straordinario, non prevedibile, di necessità e di urgenza, che impone al Governo di intervenire con uno strumento straordinario ed eccezionale qual è il decreto-legge, perché il normale *iter* legislativo non sarebbe in grado di corrispondere immediatamente a tale situazione straordinaria.

totale. Secondo la Corte, nel sindacato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza, un ruolo cruciale compete al requisito dell'omogeneità, che si atteggia come uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validità del provvedimento governativo. sostanza, la Corte afferma che, se il decreto-legge è eterogeneo e se le diverse disposizioni in esso contenute non sono riconducibili a una matrice razionalmente unitaria e non sono espressione di un disegno finalistico coerente, armonioso e unitario,

eterogeneo, è invalido e la sua invalidità non viene sanata dalla legge di conversione. La legge di conversione che converte un decreto-legge privo dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza o palesemente eterogeneo è a sua volta invalida e difatti la Corte ha dichiarato incostituzionale la legge di conversione del decreto-legge, specificando espressamente che non esiste - cito la Corte alcuna preclusione affinché la Corte stessa proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e precisamente di tipo prettamente politico, sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo ai suoi effetti. Alla luce Alla luce di questa recentissima giurisprudenza, che non è un monito, non è un *obiter*, non è una sentenza interpretativa, ma è una sentenza di accoglimento motivata in maniera chiarissima,

fa dalla senatrice Minasi, la quale ha ben spiegato che il decreto-legge contiene disposizioni che disciplinano una pluralità di materie del tutto eterogenee. Il decreto-legge, contiene disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali e disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge n. 1158 del 1971, cioè la società Stretto di Messina, contiene anche disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari; disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la laguna di Venezia; disposizioni per quanto riguarda la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari; una specifica disposizione per il Teatro di Piacenza; una disposizione specifica per il completamento di interventi strutturali; una disposizione specifica per la proroga della messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova statale Sassari-Olbia; disposizioni per la proroga di termini per l'adozione di decreti di esproprio per il completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e autostrada Cisterna-Valmontone; ma anche disposizioni per il commissariamento della piattaforma logistica intermodale del porto di Tremestieri; Tremestieri; una disposizione che specificamente disciplina l'aspettativa dei dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e poi, naturalmente, una disposizione sul Polo di alta formazione coreutica della Fondazione accademica d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala di Milano; norme sul ponte Nord di Parma; autorizzazione di spesa per la realizzazione dell'intervento della Regione Liguria a Begato (Programma innovativo per la qualità dell'abitare); disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale; norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile; misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani; naturalmente, c'è anche una disciplina del Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2; un rifinanziamento per interventi strutturali della Regione Liguria e per il completamento della Scuola politecnica Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Genova Erzelli; e poi misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internalizzazione delle imprese italiane; non potevano poi mancare, naturalmente, modifiche al codice di procedura penale (perché non c'è decreto nel quale non si intervenga anche sulla materia penale, sia quella sostanziale, sia quella procedurale); infine, una disposizione per la decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti. Onorevoli colleghi,

non sono motivate in ordine ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza, perché nel preambolo non c'è una sola parola sul perché ogni singola disposizione dovrebbe essere contenuta in un decreto-legge, ma che poi non c'è neanche alcuno alcuno sforzo argomentativo sull'omogeneità e neanche il relatore di maggioranza ha speso una parola per provare a simulare una qualche omogeneità e coerenza. concludere. GIORGIS *(PD-IDP)*. Quella che state per approvare è una legge palesemente in contrasto con i precetti costituzionali che, se la Corte dovesse dichiarare incostituzionale, come ha fatto nella sentenza che ora ho richiamato, determinerà quell'incertezza e quell'instabilità del nostro ordinamento giuridico che rappresenta un danno

significa non corrispondere all'interesse generale del Paese, e di questo dovete assumervi la responsabilità.

il decreto-legge sul quale abbiamo appena votato la questione pregiudiziale si presenta come l'ennesimo provvedimento *omnibus*, un'abnormità giuridica nella quale, con la motivazione della decretazione d'urgenza, alla fine il Governo inserisce provvedimenti di varia natura e destinazione, con la pretesa motivazione che ci sia un'urgenza che rende necessario ricorrere a questo tipo di strumento. abbiamo invitato più volte la maggioranza a rivedere questo modo di legiferare e assumersi anche le responsabilità di questa legiferazione caotica, talmente fuori fuori contesto e disordinata da avere anche impedito alla stessa maggioranza di rispettare dei termini che si era data. Penso, per esempio, al al decreto-legge che è stato posto in votazione la settimana scorsa proprio per la proroga del termine dell'adozione dei testi unici per il riordino del diritto tributario, termine non rispettato proprio perché troppi decreti-legge hanno impedito all'Assemblea e agli uffici di fare il lavoro ordinario, che poi sarebbe quello fondamentale di un Parlamento, invece di un lavoro straordinario, che dovrebbe essere episodico.

ad astenersi dal portare avanti questa prassi e soprattutto ad attenersi a un criterio di organicità e di sistematicità nella legiferazione, cioè a fare provvedimenti che abbiano un testo che riguarda un'unica materia e a non infarcirlo, come nel caso di specie, di disposizioni che riguardano autostrade, infrastrutture, investimenti strategici per il Piano Mattei, enti musicali, addirittura la proroga del termine per lo svincolo dei contratti sportivi, la modifica dei termini del processo in Cassazione e del processo penale davanti alla Corte suprema di Cassazione. Insomma, non c'è un filo conduttore. È evidentemente una miscellanea di disposizioni varie che vengono presentate con questo testo, tra l'altro alla scadenza dei lavori, prima della sospensione estiva, come se fosse la *deadline*, l'ultimo

modo, non rispetta il Parlamento questa continua e pervicace ostilità, da parte del Governo, verso le norme della libera concorrenza.

sono comunitari, perché l'Unione europea continua a ribadirli con fermezza, sanzionando e richiamando l'Italia, proprio perché la nostra legiferazione continua a violare questo principio e a fare proroghe, come nel caso delle concessioni autostradali. Prorogare i termini per i concessionari in scadenza di un ulteriore trimestre o semestre, in attesa poi di fare delle gare, cosa vuol dire? Che il regolamento dei conti relativo ai concessionari è rimandato a dicembre, perché prima c'è qualcosa che va chiarito o qualche interesse che dev'essere messo al riparo dall'eventuale gara che potrebbe esporre alla partecipazione di un concorrente non gradito? Non si capisce il motivo per il quale ci sia questa ferma ostinazione nel l'espletamento delle gare pubbliche, non diversamente da ciò che attiene alle concessioni balneari e portuali, un tema nel quale l'Italia continua a essere assolutamente inadempiente ai princìpi comunitari.

applica e dispone ogni volta in cui è necessario, secondo le sue previsioni, accelerare i tempi per la realizzazione di un'opera, fare una sorta di resoconto di ciò che è stato fatto comunque pacificare gli animi e trasmettere un messaggio di sicurezza e di tranquillità: non vi preoccupate, sta arrivando il commissario straordinario. E allora accade anche l'incredibile, cioè che nello stesso testo, da un lato, inserite una disposizione con la quale

portuale di Tremestieri, nella città di Messina. Quindi con l'articolo precedente li riducete, o almeno dite che bisogna riorganizzarli e ridurli, e in quello successivo ne nominate uno nuovo. *(Applausi)*. Francamente, siete stupefacenti in questa vostra tecnica legislativa. Per quanto riguarda la nomina del commissario straordinario per il porto di Tremestieri, mi corre l'obbligo di esprimere sicuramente un apprezzamento al Governo per essersi interessato a quest'opera, che nasce con i fondi straordinari dell'emergenza traffico per la città di Messina, che è città di frontiera che subisce l'attraversamento del traffico pesante che la intasa e la blocca, quindi ha sicuramente bisogno ancor prima della realizzazione del ponte, di un porto per il traffico pesante, opera che per varie vicissitudini si era arenata e che poi, anche a causa della crisi delle materie prime e della crisi congiunturale economica, con la dotazione economica già esistente non sarebbe stato possibile realizzare. Ben venga, quindi, il finanziamento che è stato trovato

dire sempre che si vuole ricorrere alla nomina di un commissario e poi però, anche quando la finalità può essere condivisa, sganciare tale nomina da una verifica

il quale avevamo chiesto semplicemente il rispetto dei criteri legali, ossia che il commissario venisse scelto fra persone di comprovata esperienza e competenza nel settore dei servizi portuali, nell'ambito di un elenco di tecnici individuati e approvati dalle Commissioni parlamentari competenti e poi nominato con un decreto a firma congiunta dai Presidenti di Camera e Senato, per restituire al Parlamento il ruolo principale. Vogliamo nominare un commissario? Non facciamo come abbiamo fatto per il commissario del PNRR o per quello contro gli insediamenti abitativi del caporalato. Non nominiamo l'ennesimo prefetto, che poi si trova a gestire un'opera per la quale non ha competenze tecniche e non ha uffici tecnici che lo possano supportare Nominiamo persone competenti, ci può anche stare, ma ridiamo centralità e controllo al Parlamento, cosa che ancora una volta in questo testo non si vede. Il Parlamento viene nuovamente esautorato dalla scelta che a questo punto è appannaggio esclusivo del Governo che - a prescindere da come deciderà e su chi ricadrà la sua preferenza - certamente non potrà darci nessuna spiegazione in termini di trasparenza e di capacità di scelta, ma probabilmente si ispirerà ad altri criteri.

sua eterogeneità, vorrei segnalare che un emendamento approvato alla Camera dei deputati prevede la possibilità per il personale dipendente a tempo indeterminato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di fruire dell'aspettativa e avviare o dell'aspettativa e avviare o proseguire nell'attività professionale o imprenditoriale. A me risultava che il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione fosse esclusivo e che quindi non ci fosse la possibilità di utilizzare l'aspettativa

C'è stata una lunga discussione un anno fa, quando il Governo si è insediato e ci ha comunicato che il Paese non si poteva permettere di spendere 7 miliardi per il reddito di cittadinanza, perché era necessario fare altro. Secondo voi, il Mezzogiorno d'Italia ha più bisogno del Ponte o di un reddito per affrontare i problemi della povertà e quindi intervenire sull'inclusione?

di fronte ai cambiamenti climatici è sempre peggiore. I commissari straordinari sono appunto tali e, nel momento in cui si crea una struttura come l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con i compiti di coordinamento della loro attività e monitoraggio sulla realizzazione delle opere commissariate, forse non vi rendete conto che bisogna decidere cosa fare,

Come tutti sappiamo, i commissari hanno poteri straordinari, quindi continuano ad andare in questa direzione, mettendo in discussione anche il compito delle autonomie locali.

questo Governo e questi continui decreti-legge dove vogliano andare. Cercavo di darmi una risposta concreta, sostanziale, anche argomentata e l'ho trovata, come sempre, nella letteratura. Ebbene sì, secondo me, questo Governo ha la velleità di andare

di disorientare lo spettatore con dialoghi illogici e con scelte di illogica relazione. Ecco, trovo che nelle ultime settimane e negli ultimi mesi ci sia una sorta di volontà di disorientare i cittadini. Questi decreti-legge continui e soprattutto che sembrano in contrasto con la realtà mi sanno tanto di teatro dell'assurdo. Mi spiego meglio.

siamo praticamente al collasso dei trasporti. Io vengo dalla Sicilia e per delle settimane ho avuto difficoltà a raggiungere Roma, perché la tratta Villa San Giovanni-Roma era proprio interrotta. Nel mio territorio facciamo fatica - ebbene sì - ad utilizzare l'acqua, perché per diverse ore durante il giorno non c'è. non c'è. Sapete dove non c'è? A Messina, dove si vuole praticamente iniziare un cantiere che sarà lungo 18 chilometri. Allora, in questa realtà

di come non fare brutta figura con i cittadini, ai quali aveva detto: cominciamo i cantieri oggi, anzi domani, prima dell'estate o alla fine dell'estate. Siccome non può tenere testa alle sue promesse, fatte fondamentalmente a se stesso, perché non gli crede più nessuno, che cosa fa in questo decreto delle infrastrutture, atto secondo? L'irreale: addirittura seziona il progetto per poterlo approvare a pezzi. Signori, guardate che se il primo atto è quello della realtà che vediamo tutti, che vediamo noi cittadini, di un'Italia al collasso, l'atto secondo è quello di un Governo che invece racconta un Paese perfetto, che può sognare un ponte che però non sa fare, allora si inventa di farlo a pezzi; una Presidente del Consiglio che praticamente continua a fare la *leader* di opposizione e si racconta e dice quanto è brava e bella (meno male che se lo dice da sola), elogiando il famoso PNRR, che neanche ha votato e che non avrebbe voluto. *(Applausi)*. Ecco, se noi fossimo intellettualmente disonesti, come lo sono stati quelli che adesso sono in maggioranza e all'epoca, quando noi governavamo, erano all'opposizione, chiederemmo le dimissioni di Salvini immediatamente. Solo che intellettualmente siamo onesti e sappiamo che tutta la devastazione non può essere in capo soltanto a un Ministro, che però avrebbe la responsabilità di occuparsi dei problemi dei trasporti e non di spostare l'attenzione. Oggi ero in treno e cercavo di sbirciare nelle sue pagine Facebook; sì, perché

teatro dell'assurdo? La situazione è drammatica, lui se ne infischia e potremmo anche tutto sommato resistere. No, peggiora la situazione. Come la peggiora? Con questo decreto-legge - vado a elencare prevedete l'approvazione del progetto esecutivo, come dicevo prima, per fasi, a pezzettini; non sappiamo se il ponte lo facciamo, non sappiamo se ci sono le risorse per tutto e non sappiamo se il progetto definitivo sarà cantierabile, ma intanto vi mettiamo un pilone qua e una rampa là, così facciamo vedere che muoviamo i cantieri *(Applausi)*, solo per farsi la famosa foto con la ruspa. Non prevedete - gravissimo, a nostro avviso - un un termine: siccome quello che avevate previsto non lo potete soddisfare, lo avete tolto. È così: ma sì, che Messina sia un cantiere infinito e anche Villa San Giovanni e anche mezza Sicilia; cosa vi importa, purché si possa dire che avete cominciato, per finta, i lavori del ponte? Attenzione, oltre al danno, la beffa: la certificazione delle spese - udite, udite - non la fa un ente terzo; assolutamente no. Chi la fa? Un consulente nominato da Salvini. Ma vi sembra trasparenza? Vi sembra corretto procedere in questo modo con i soldi dei contribuenti? A proposito di soldi: ma sì, siccome nell'immaginario di questo Governo tutto ha un prezzo, ma pochissime cose hanno un valore, aumentiamo i soldi per comprare quei terreni e permettere alle persone di andare via più facilmente, tanto i soldi sono di tutti i cittadini. Purché voi possiate cominciare i cantieri, cantieri, buttiamo i soldi così. Attenzione, signori, perché il Paese non è in vendita, non tutto ha un prezzo e non tutto è in vendita. A proposito di prezzi, di costi e quant'altro, ricordiamoci che nelle pagine e pagine di questo progetto, che ancora dev'essere completato, ha parti manchevoli e quant'altro, non c'è un solo elaborato di stima dei costi. Ma come si fa? Adesso voi avete vinto le elezioni e volete fare il ponte: il diritto, ma non avete il diritto di prendere in giro i cittadini. Voi potete fare un ponte, ma quando sarete in grado di farlo, scegliete di farlo con un progetto completo e con le risorse in tasca, perché il diritto di governare non comprende quello di prendere in giro i cittadini. *(Applausi)*. E ancora, la società Stretto di Messina è in perdita di 80 milioni nell'ultimo bilancio del 2023. Com'è che, nonostante questo, continua ad assumere dipendenti e consulenti? Com'è possibile? Penso che i cittadini

sia un decretino. A volte l'italiano è come se anticipasse, nella terminologia, la sostanza dei decreti. Fate così tanti decretini che, secondo me, nella loro sostanza sono poverini. *(Applausi)*. Se non fosse che sono anche pericolosi, potremmo anche ridere, come ho riso quando un sottosegretario della Lega è venuto a Messina nella Zona Falcata con l'elicottero. Signori miei, anche io sono stata Sottosegretaria: ora, non perché sono del MoVimento 5 Stelle, ma mi sono mossa in taxi. Non è che per arrivare nella Zona Falcata servisse l'elicottero. Questo per raccontare un po' anche la sostanza. Evidentemente, il ponte lo fanno per questi Sottosegretari, che sennò devono prendere gli elicotteri per arrivare a Messina; forse è meglio Detto questo, il teatro dell'assurdo: reale, atto primo; irreale, atto secondo; incubo, atto terzo, con questi decreti assurdi. Se non fosse non fosse davvero - perché io amo la letteratura - anche la fase del teatro dell'assurdo, credo che forse sarebbe il caso che su questo Governo calasse il sipario.

probabilmente lascia in salute e noi siamo orgogliosi che anche il ministro Salvini, che rimarrà per molti anni in quel Ministero, porterà avanti in salute tutte le opere

curiosamente a porre dei dubbi circa il metodo e la matrice unitaria del contenuto di questi decreti, farò

continuare con tantissimi altri precedessori. Ebbene, adesso, in una visione unitaria, che la politica del centrodestra ha inteso portare nella guida del Paese, siamo consci - e ribadisco siamo sempre orgogliosamente - del fatto che questo Governo nei suoi decreti ha posto delle precise linee guida, che andrò brevemente ad esporre. Si parlava del Ponte sullo Stretto, cui sono state portate tante critiche. Il fatto di procedere per fasi costruttive,

procedendo *step by step* nella realizzazione del ponte. Ciò ben sapendo che nel corso del tempo, anche a causa dell'instabilità geopolitica e di tutto quello che abbiamo subito con la pandemia e di ciò che è avvenuto dopo, può determinare una variazione dei costi, sui quali l'interezza progettuale di un'opera di queste dimensioni potrebbe comportare una difficoltà gestionale nel momento in cui si dovessero manifestare

delle discariche ai commissari straordinari che si occupano di tante materie. In questo caso ci occupiamo di quelli che stanno portando avanti delle opere indispensabili per il nostro Paese. Stiamo cercando di riordinare funzioni quali i commissari sono assolutamente ligi e che vedono in queste figure la soluzione, in via ovviamente derogatoria di norme che sarebbero pletoriche per la rapida esecuzione di interventi strategici. Siamo di fronte all'applicazione di un metodo, quello dei commissari, che sta lentamente, ma in maniera evidente e con molta praticità,

di importanza strategica sia per il fatto di attraversare una base militare come Camp Darby, ma soprattutto per i nuovi

da ora in poi sarà realizzata attraverso un adeguamento stradale da ANAS. Ebbene, su quella strada, sulla quale purtroppo ha trovato la morte

del Governo Renzi e poi per una serie di errori che si sono accumulati con i provvedimenti varati nel 2019 e nel 2021. È stata posta una precisa condizione per avere perlomeno un metodo di quantificazione del costo dell'acquisto dei progetti già realizzati Società autostrada tirrenica, per poter così cantierare finalmente i vari lotti che recentemente, anche da parte di chi governa la Regione Toscana, in maniera molto confusa si è cercato di finanziare addirittura cercando di proporre alla *premier* Meloni di inserire 100 milioni su questa opera, per la quale peraltro in gran parte non sono ancora stati completati gli stati progettuali dai quali

ci sono 20 milioni destinati in contabilità al Commissario straordinario per la realizzazione della base militare dei reparti speciali dei gruppi di intervento speciale Tuscania dei Carabinieri paracadutisti. Si tratta di un'opera attesissima, che permetterà di recuperare un sito che è già nella disponibilità del Ministero della difesa, ma che renderà finalmente un minimo di dignità ai reparti più conosciuti e più noti a livello internazionale, dei quali abbiamo un elenco di missioni e di operazioni che

ostacolare anche la realizzazione di quest'opera, adducendo ragioni assolutamente assurde rispetto alle quali spero che la concretezza

studi per le applicazioni militari sarà il sito nel quale sul territorio di Pisa verrà realizzata questa grande opera. In conclusione, questo è un provvedimento strategico che modernizza e potenzia gli investimenti nel nostro Paese, è un passo decisivo verso una maggiore trasparenza ed efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici, con opere finalizzate a migliorare la connettività e la sicurezza dei trasporti, la transizione ecologica, la digitalizzazione e l'innovazione. E naturalmente queste misure avranno un impatto positivo di lungo termine sullo sviluppo del Paese.

prassi che, nell'occasione del provvedimento in discussione, è certamente aggravata da un livello di pluralità delle materie trattate senza dubbio elusivo del dettato costituzionale, della giurisprudenza costituzionale che puntualmente ignorate e che non avvertite più la sensibilità né il pudore istituzionale di dover giustificare in qualche misura. Il senatore Giorgis prima lo ha detto molto meglio di come possa dirlo io adesso. E pensare che nel corso di un'estate così gravemente caratterizzata da problemi importanti nel settore dei trasporti e da un fenomeno della siccità tanto drammatico, la scelta del Governo di intervenire con un provvedimento necessario e urgente sarebbe persino potuta essere, per una volta, una buona notizia, ma siamo al paradosso, per chi ci guarda, che magari pensa che stiamo discutendo di ciò che è davvero urgente e indifferibile: noi discutiamo di tutto tranne che di quello che per l'interesse di questo Paese è davvero urgente e indifferibile. Purtroppo basta leggere il testo del decreto in conversione per capire come delle questioni necessarie e urgenti non vi sia alcuna traccia, per favorire tutt'altre materie e urgenze, in particolare quelle ritenute tali dalla Lega, in una dialettica interna con Fratelli d'Italia e Forza Italia sempre più incontenibile. Diciamo la verità: la Lega, ancora una volta, anche su questo decreto-legge, l'ha fatta da padrona ed è riuscita in quello che da più parti è stato definito un assalto alla diligenza, raccogliendo una notevole quantità di risorse per i territori di proprio interesse a solo fine elettorale e di consenso e il palese nervosismo dei partiti di Governo è il più chiaro segnale di questa dinamica. *(Applausi)*. Nel dibattito alla Camera, i colleghi del Partito Democratico lo hanno definito un provvedimento emblema del salvinismo che, insieme al decreto casa, dimostra chi davvero guida il Governo con buona pace della presidente Meloni. E basta analizzare nel merito le norme contenute nel provvedimento in discussione per capirne la genesi politica e i veri obiettivi. Penso, ad esempio, a quanto viene stabilito all'articolo 1 in materia di concessioni autostradali. Su quelle in scadenza a fine anno abbiamo cercato, con alcuni emendamenti, di proporre che il recupero dei finanziamenti delle opere per i concessionari avvenga per la durata media di vita dell'opera, consentendo così di avere un impatto minore sui pedaggi pagati da chi percorre queste strade. Una proposta a tutela dei cittadini utenti, ma che, nonostante il suo contenuto del tutto ragionevole, è stata bocciata; una proposta che ci risulta peraltro essere al vaglio del Governo su provvedimenti in arrivo in Parlamento. in particolare, all'annunciato disegno di legge sulla concorrenza, che del tema delle concessioni autostradali si occuperà ampiamente e che ha già subìto pesanti critiche dalla Commissione europea e dall'Autorità per i trasporti, sui due temi del rischio traffico e del pedaggio unico, che a quanto pare sarebbero trasferiti allo Stato, ancora una volta secondo gli indiscutibili *desiderata* del ministro Salvini. Decisamente emblematico del decreto-legge in discussione è l'articolo 2, l'articolo dedicato al Ponte sullo Stretto: un insieme di procedure in deroga per accelerare l'*iter* tecnico ed amministrativo, sacrificando i principi di trasparenza e buona amministrazione sull'altare della propaganda di Governo. Abbiamo rimarcato, nel dibattito in Aula e nelle Commissioni, tutta la nostra contrarietà a questa opera costosa e dannosa, anche avanzando specifici emendamenti, tutti puntualmente ignorati. Insieme ai nostri emendamenti, circostanza certamente più grave: avete ignorato anche i pareri del CIPESS e del Consiglio di Stato, nonché il fatto che la valutazione di impatto ambientale è ancora in corso e ogni decisione in merito ad eventuali modalità di realizzazione dell'opera per lotti funzionali andrebbe rinviata all'esito dell'*iter* autorizzativo autorizzativo della VIA, per il quale sono state richieste integrazioni all'originario progetto, senza le quali la Commissione non è in condizione di decidere. Le medesime integrazioni, peraltro, che furono oggetto di analoga richiesta della VIA ben nove anni fa e che a tutt'oggi non sono state superate. Faccio riferimento, in particolare, alle questioni riguardanti la sicurezza sismica dell'opera, ma molto altro si potrebbe dire sulla incompatibilità delle procedure di affidamento con la normativa europea in materia di incarichi diretti, già segnalate dall'ANAC; come anche sul contrasto con la normativa in materia di piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, nonché sull'annosa questione degli espropri. Su tale questione il decreto in conversione ritorna ancora una volta e lo fa introducendo una sorta di procedura *ad hoc* per il Ponte sullo Stretto, che rappresenta un assoluto precedente rispetto alle ordinarie procedure di esproprio in materia di opere pubbliche, prevedendo, tra le altre cose, un tetto massimo di 40 milioni. Ma senza un progetto esecutivo, da dove viene questa cifra? E per tutti coloro che dovessero ritrovarsi fuori, una volta raggiunto questo arbitrario limite massimo, in che modo si procederà a ristorare gli eventuali espropri? Scelte politiche e soluzioni normative del tutto fuori dalla logica, proprio mentre le Regioni toccate da questa faraonica opera soffrono gravemente per una siccità che sta mettendo in ginocchio le reti idriche, l'agricoltura, i trasporti, l'economia: questi sì, settori che avrebbero bisogno delle risorse pubbliche bruciate per il Ponte, al fine di vedere mitigati i disagi che i cittadini del Mezzogiorno, e non solo, soffrono da decenni. Dove sono gli interventi necessari per far fronte alla storica siccità che vive il Paese? Penso a tutti quei progetti del PNRR rimasti nei cassetti oppure ancora in attesa di essere dotati delle rispettive risorse. Ma faccio riferimento anche al lavoro svolto dal commissario straordinario per la siccità, che ha individuato ventisette interventi solo per la Sicilia, con investimenti pari a 830 milioni di euro, che però non sono stati finanziati. È una situazione grave, che purtroppo non è esclusiva della Sicilia. signor Presidente, alla mia terra, il Fucino, orto verde d'Abruzzo, che vive una delle situazioni più complesse della sua storia, con il razionamento delle acque per l'irrigazione dei campi. Una condizione paradossale dovuta a scelte politiche chiare, delle quali in passato abbiamo a più riprese interessato il Governo e anche quest'Aula. La Regione, governata dalla destra da oltre cinque anni, ha tagliato 50 milioni stanziati dalla Giunta di centrosinistra nel 2014 per la realizzazione di un impianto irriguo, che oggi ci avrebbe consentito di affrontare la situazione con ben altri strumenti. Non saremmo oggi spettatori indignati delle difficoltà delle imprese agricole, dei canali in secca, della fauna ittica sui bordi dei fossati, delle difficoltà di tanti amministratori e amministratrici locali. Cinquanta milioni tagliati per finanziare sagre e polisportive e mai più ripristinati, nonostante le promesse. Un chiaro esempio della modalità con cui questa destra governa nel Paese e sui territori. Tornando al provvedimento e a quanto prevede l'articolo 3, in materia di gestioni commissariali, avremmo voluto esprimerci anche noi a favore, se si fosse aperto un dialogo effettivo in Parlamento. Siamo anche noi, infatti, persuasi che una razionalizzazione delle materie, come indicato anche dall'ANAC, sia auspicabile, in particolare per un Governo che, come ricordava il collega Simiani alla Camera, ha stabilito un *record*, con la nomina di ben sessanta commissari sulle più disparate questioni. D'altra parte, senatore Potenti, lei giustamente ha appena rivendicato che questo è un metodo: la via commissariale al Governo, del tutto coerente con l'idea di fare della decretazione d'urgenza uno strumento ordinario. Ma è un nominificio, esattamente in linea con quanto previsto nel decreto in materia di CCS. All'articolo 6, si stabilisce la nascita di un Comitato per la gestione e lo sviluppo di questa tecnologia di recupero della CO2, una tecnologia non in linea con la direttiva europea ATS e non coerente con il principio che chi inquina paga. Nel caso in discussione, infatti, le risorse derivate dalle aste per la CO2 servirebbero semplicemente per pagare gli emolumenti dei componenti del nascente comitato. In ultima analisi e pur volendo sempre rinunciare a pre-giudizi, siamo di fronte alla conversione di un decreto che sui temi infrastrutturali non si cura delle autentiche criticità del Paese, non guarda alla programmazione, non interviene sulle emergenze, né sui temi ambientali e sulla prevenzione dei cambiamenti climatici; non mette in campo misure e risorse, ma si limita a guardare al passato. Sul Ponte sullo Stretto, sport e norme ordinamentali, nella migliore delle ipotesi alimenta confusione, nella peggiore genera numerose forzature: una modalità di governare e legiferare coerente con la prassi di questo Governo. Con altrettanta coerenza non possiamo noi che ritenerci insoddisfatti e giudicare questo decreto-legge su materie tanto strategiche l'ennesima occasione persa per il Governo, persa per il Parlamento e in ultima istanza persa per il Paese.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1206, di conversione, con

apre una nuova finestra"). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 89, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

vivere in quest'Aula un'esperienza un po' tardiva ma ancora entusiasta, e non tanto per stare con senatori amici e amiche che più o meno la pensano come me, anche se rifiutiamo un pochino l'omogeneità del sapere e delle idee, ma perché da sempre cerco di essere stimolato a pensare e a pensare meglio dall'opposizione. Purtroppo, in quest'ultimo periodo mi rattristo molto perché non sento dalle opposizioni stimolazioni di alcun tipo. Sento solamente delegittimazione, mancanza di proposte, derisione, poca cultura politica. Non si offendano per questo. Qualcuno dirà che non colgo le stimolazioni perché sono anziano. Forse non coglierò certe sensazioni stimolanti, ma ancora penso di averle. Credo che la politica sia fatta soprattutto di proposte e di controproposte, mai di delegittimazione dell'avversario anche in maniera un po' rozza e un po' crudele, ma senza substrato reale. Ho colto con piacere il colto intervento della senatrice Floridia, il teatro dell'assurdo, che mi dà agio di utilizzare questo messaggio per parlare della musica. In una chiesa qui vicino si è inventata la Tosca, recondita armonia di colori diversi. Bene, il provvedimento di oggi, non ha nulla di recondito, ma armonie che compongono frasi politiche, provvedimenti interni che hanno un punto in comune, una grande armonia per raggiungere un obiettivo: il benessere del cittadino italiano. Questo è quello che ci deve interessare. Ministro Ministro Ciriani, ci mancherebbe altro, esprimeremo un voto favorevole alla fiducia più di altre volte perché è anche frutto di un pensiero complesso per ognuno di noi. Abbiamo superato momenti di difficile interpretazione perché quando il decreto-legge è *omnibus* ricomporre l'armonia non è sempre facile in questa società che va così in fretta anche al nostro interno. C'è un punto. Qualcuno dice che bisogna restituire centralità al Senato e al Parlamento. Più centralità di così? Avete, come sempre, tutte le possibilità di manifestare certamente dissenso - ci mancherebbe - ma anche proposte che però non ascolto. E allora cosa consegneremo alla storia? Un teatro armonico e non da incubo, un coro possibilmente con poche stonature, ma soprattutto tanto, tanto entusiasmo di voler cambiare le cose, trovando una resistenza incomprensibile da parte dell'opposizione. Sono stato una vita all'opposizione e non ho quasi mai cercato di fare la "cianchetta" gambe, cercando di superarli anche in coerenza con quanto è stato detto nella proposta e non nella protesta. Scusate il riferimento autobiografico; ieri a Chianciano ho visto una nipotina,

tesi verso l'ascolto di quello che vede. Non dico ascolto per quello che vede, è una sintesi delle percezioni. Cosa comprenderà tra qualche anno del gioco della democrazia tra maggioranza e opposizione? Potrà vedere i lati positivi di questa cosa che, ripeto, si chiama il gioco importantissimo, decisivo, della democrazia o coglierà da una parte persone che propongono, magari con qualche errore, e dall'altra parte gente che è solo pronta alla ghigliottina alla ghigliottina e alla fucilazione preventiva? Io spero che Viola non sappia quello che sta accadendo e spero che veda quanto di buono in comune, anche nelle differenze e nelle diverse opinioni, si possa avere. Un decreto-legge *omnibus* complesso deve unire, non dividere, soprattutto con proposte che completano oppure alternative, ma non con abbai di odio, di discriminazione e di preventiva suggestione negativa, perché questa non è democrazia, ma è opposizione opposizione - scusatemi se lo dico - acefala, e un pochino di cervello me ne intendo, anche se ne ho ancora pochino. Quindi, sinceramente, con tutto il cuore, i giovani ma anche i meno giovani (mi ci metto pure io), anche nella difficile realtà di costruire un tessuto comprensibile, di fare un coro senza tante stonature, anzi armonico, perché su questo vive la democrazia, con chi ha il coraggio di cambiare e chi ha solo la paura e il *pavor* che qualcuno cambi qualcosa, perché preferisce che le cose non cambino mai. *(Applausi)*.

francamente - Presidente, lo dico per suo tramite - non ho davvero capito che cosa ravvisasse all'interno di questo provvedimento (anche chiamarlo *omnibus* è già una concessione enorme in termini di credibilità), in riferimento al presunto cambiamento che il Paese dovrebbe fare. Provo a spiegarmi in pochissime coordinate. In questo provvedimento ci sono degli interventi, direi del tutto marginali e non risolutivi, di varia natura e di vario genere. Poi c'è sempre una straordinaria attenzione a Genova, e questo va riconosciuto: su un decreto complessivo, ci sono sempre tre o quattro interventi che riguardano Genova, alcuni sensati, alcuni meno sensati, alcuni risolutivi, alcuni meno risolutivi, come segnale del fatto che dentro il Ministero c'è chi si occupa di Genova. Questo l'abbiamo capito ed io personalmente lo apprezzo, altri magari no. Però la visione dentro questo il fatto stesso di chiamarlo decreto-legge infrastrutture è francamente sbalorditivo e vi spiego perché. È sbalorditivo perché abbiamo dei problemi oggettivi che sono la causa di quello che sta accadendo nel Paese. I ritardi dei treni non sono frutto del destino cinico e baro. Perché si stanno configurando ora? Perché la nostra linea sta collassando. Quella dell'Alta velocità, realizzata circa trent'anni fa, ha dei requisiti tecnici, soprattutto nella tratta Firenze-Roma, che creano dei colli di bottiglia, cioè i parametri per i 300 chilometri orari o similari

ulteriormente a creare un problema nel momento in cui c'è un sovraccarico di treni e un sovraccarico di offerta. Quindi, è una rete inadeguata rispetto a una serie di servizi che devono essere ulteriormente implementati per un Paese che - scusate se è poco - è l'emblema della potenzialità delle opportunità turistiche, l'emblema della logistica

e quindi ci vogliono investimenti di manutenzione, di adeguamento e di potenziamento, che cosa si fa nel PNRR? Si tagliano - vado in sequenza le linee di collegamento con l'Europa del Nord (Verona-Brennero); le connessioni diagonali della Roma-Pescara e parzialmente i collegamenti ferroviari dell'Alta velocità Napoli-Bari; i collegamenti ferroviari della Palermo-Catania-Messina; le connessioni diagonali della Orte-Falconara; le connessioni diagonali della Taranto-Metaponto-Potenza; il sistema ferroviario della

milioni di tagli. Poi, andiamo avanti, perché ci sono anche i tagli alle stazioni ferroviarie del Sud. Chiunque vada al Sud, naturalmente oggi trova delle stazioni ferroviarie meravigliose, che non hanno bisogno di quegli investimenti. Sono stati fatti 300 milioni di tagli sulle stazioni. Perché si sono tagliate queste risorse? Perché il Ministero delle infrastrutture, guidato da Salvini, non riesce a spendere queste risorse. Secondo l'audizione della senatrice Paita, qual è il Ministero che ha speso peggio le risorse sul PNRR, anzi che non ha proprio speso le risorse sul PNRR? Il premio va a Salvini: di spesa. Però, vedete, la differenza rispetto agli altri Ministeri - vi invito a questo ragionamento - è la seguente:

Se volete avere un parametro rispetto all'incapacità di governare e programmare il PNRR, dovete guardare in faccia Salvini *(Applausi)*, perché mentre in tutti gli altri casi può trovare una scusa, una responsabilità in un povero ente locale che magari ha un solo dipendente o due dipendenti e non riesce a fare quella gara, nel caso della rete ferroviaria il Ministero dà, il Ministero deve rispondere e le responsabilità sono in capo a un unico soggetto, che guarda caso è Salvini, il quale non vede quello che sta succedendo nel Paese. Il ministro Salvini va a fare il video alle stazioni dei taxi nell'unico giorno in cui ci sono i taxi; non so se li ha chiamati lui, non mi permetto di dirlo, però chiunque di noi, non solo cittadini, ma anche parlamentari, abbia avuto bisogno di un taxi in questi mesi, ha avuto l'amara sorpresa di un sistema che non c'è, di una risposta che non c'è. Se questa risposta non c'è in una città come Roma, dove il trasporto pubblico è totalmente inadeguato, non solo per responsabilità di Salvini, ma diciamo che da quando c'è lui non è che siano cambiate tanto le cose, allora c'è un problema grosso che significa sicurezza dei cittadini, che non sanno come muoversi, che significa impossibilità di dare opportunità ai nostri ragazzi, che non hanno a disposizione nulla; in alcuni casi non hanno l'Alta velocità, in altri casi non hanno le metropolitane, in altri casi non hanno nemmeno i taxi. Di fronte a tutto questo scenario lui non vede il problema e casualmente va a prendere il taxi il giorno in cui il taxi c'è. è per il Paese una vera e propria presa per i fondelli. A fronte di questo scenario apocalittico che vi ho descritto, con la rete dell'alta velocità che sta collassando e i sistemi regionali che non stanno andando avanti, cosa si mette in campo? Un decreto che non risolve niente, quello di oggi. E però ce n'è uno che sta per arrivare e di questo voglio parlarvi negli ultimi minuti che ho a disposizione: si tratta del provvedimento sulla concorrenza. Lì la strategia è davvero incredibile. Voi sapete che un altro dei problemi di questo Paese è quello dell'adeguamento, della manutenzione e della realizzazione di nuove autostrade, che non c'entrano con il PNRR, perché non possono essere finanziate con il PNRR. C'entrano con cosa? Con la strategia che noi abbiamo, cioè concessioni per le autostrade date dal Ministero e quindi il controllo del Ministero sugli adeguamenti. Purtroppo chi vi parla è esponente di una Regione che, a causa del cattivo funzionamento tra il potere di controllo del Ministero e le manutenzioni in termini di sicurezza delle autostrade, ha avuto il dispiacere

il simbolo del degrado di un Paese e verso le quali va, ancora una volta, tutta la nostra riconoscenza e tutto il nostro pensiero.

sanare i debiti delle concessioni autostradali del Nord (cioè esattamente l'opposto dell'autonomia), della Pedemontana veneta e di tante altre di questo tipo, perché questo aveva in mente ; l'altra va invece a realizzare nuovi investimenti. Ora, se tu hai dieci e dividi per due, come fai, se già oggi non hai le risorse per realizzare nuovi investimenti? Chiudo, Presidente. Per fortuna questa strategia, un po' perché l'Europa gli ha detto che non si poteva fare e un po' perché forse anche a qualcun altro sarà venuto in mente che era una vera e propria follia, pare che stia rientrando. Ma il tentativo c'era e sapete cosa significa questa cosa? L'autonomia al contrario. Prima si dà una funzione fondamentale come quella delle autostrade a Regioni che non sono in grado di portarla avanti e poi, quando le cose non funzionano, si creano i debiti e non si riescono a fare gli investimenti, allora si chiamano a raccolta tutti i cittadini italiani per compensare quei debiti e per realizzare gli investimenti. *(Applausi)*. Ecco perché voi avete un'idea sbagliata sull'autonomia; ce l'avete su questo e ce l'avete sui porti. Voi pensate che il Paese si possa dividere in mille pezzi, perché tanto poi la responsabilità la pagheranno tutti,

Aspetti, perché, se lei parla senza microfono, non si sente niente. Chiudo dicendo che le infrastrutture servono a sviluppare un Paese e, se tu hai un Ministro come Salvini, ti puoi scordare di riuscire a muoverti, ma anche di sviluppare un Paese.

sul merito di alcune questioni. Abbiamo criticato e continuiamo a criticare come opposizione (io credo giustamente) l'uso dei decreti-legge. Ora, però, devo dire che questa maggioranza

vorrei sottolineare che non c'era alcun intervento sul caporalato e che questo è stato inserito poi successivamente, con un emendamento del Governo. Quindi non se ne erano è accorti. Ora stiamo parlando di una situazione di emergenza e io credo che una delle emergenze più gravi

Noi stiamo discutendo di fare un ponte a pezzetti - e anche questa è una bella novità, e noi speriamo

il cittadino normale non può farlo e si deve adeguare a una situazione nella quale il ritardo è una

Discutiamo di infrastrutture che servono al Paese? Discutiamo di infrastrutture che servono alla Calabria e alla Sicilia, dove

c'è un accordo tra la più grande impresa nell'agroindustria italiana e il Ministero dell'agricoltura algerino per coltivazioni su 36.000 ettari. Abbiamo sentito tutti che neanche un chicco di grano arriverà in Italia, perché quelle risorse devono rimanere dove si investe;

voglio sottolineare che si realizzano queste cose utilizzando i soldi che erano destinati agli interventi sul clima, e cioè 4 miliardi si spostano da un'altra parte.

il Governo è intervenuto su questo decreto-legge per velocizzare le procedure di alcune opere pubbliche ritenute strategiche e la *governance* dei gestori di alcune infrastrutture, come le autostrade. Sono inoltre previste altre disposizioni per velocizzare la realizzazione di alcune opere molto attese nel nostro Paese: innanzitutto per accelerare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un'opera strategica la cui realizzazione è considerata un punto di svolta nel nostro sistema infrastrutturale sin dai tempi dei Governi Berlusconi; un'opera che avrà ricadute enormi sul territorio per i molti anni previsti per la realizzazione e, una volta completata, cambierà totalmente l'economia delle due Regioni interessate, rendendole un *hub* fondamentale di collegamento dall'Europa verso il Mediterraneo. L'intervento normativo in esame risolve una serie di criticità e amplia il margine di manovra sugli aumenti dei costi in corso d'opera. Vengono altresì riviste le procedure di esproprio, prevedendo che vengano tutelati sia gli operatori economici coinvolti nella realizzazione dell'opera, sia i proprietari che oggi risiedono nei territori interessati. Coniugare l'interesse pubblico a realizzare un'opera strategica e tanti interessi dei residenti sulle aree in cui l'opera deve essere realizzata è un punto fermo. Quanto fatto a Genova, dopo il crollo del Ponte Morandi, con la successiva ricostruzione, ha riproposto il tema della procedura della cessione volontaria al posto delle espropriazioni forzate. Come ho già detto molte volte in quest'Aula, le persone vanno convinte e non obbligate. Gli immobili interessati avranno quindi una valutazione ulteriore, che va oltre quella di mercato, potendo contare su un'indennità aggiuntiva a favore dei proprietari che dovranno ricollocarsi. Ma non c'è solo il Ponte in questo decreto-legge. Sono previste anche una razionalizzazione dei compiti e le funzioni dei commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari. Sono più di cento gli interventi interessati da disposizioni, che interessano porti, dighe, reti ferroviarie, strade, edilizia stradale. commissari che si occupano di queste opere saranno interessati da un intervento di razionalizzazione, che sarà realizzato attraverso un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Così come verranno individuate le opere e i progetti che riguardano la realizzazione della rete dei trasporti transeuropea. L'Europa deve diventare sempre più un'Unione che abbia collegamenti efficienti e veloci tra i diversi Paesi e l'Italia deve essere centrale in questi collegamenti strategici. Ci sono tempi da rispettare per raggiungere gli obiettivi previsti: completare entro il 2030 la rete centrale ed entro il 2050 la rete globale. Allo scopo di contribuire all'integrazione multimodale delle infrastrutture di trasporto dell'Unione europea, saranno quindi privilegiati i collegamenti transfrontalieri. Diverse altre sono le opere interessate dalle disposizioni, che ne velocizzano la realizzazione. Ad esempio, sull'autostrada Cisterna-Valmontone vengono accelerate le procedure di realizzazione, a fronte di quasi 400 milioni di euro stanziati da utilizzare nel periodo dal 2024 al 2034. Tra le altre opere interessate all'intervento in esame, c'è la parte toscana della Tirrenica, con la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento della tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi, regolamentando il passaggio dall'attuale società concessionaria all'ANAS. Tra gli altri interventi che meritano particolare menzione c'è quello che riguarda la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico di Peschiera, per il quale verranno previste ulteriori risorse al fine di garantire un'adeguata fornitura di acqua alla Capitale, che il prossimo anno sarà interessata da un evento straordinario, il Giubileo, un evento per il quale è previsto l'arrivo di circa trenta milioni di pellegrini. inoltre, interventi con opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica per la funzionalità infrastrutturale sulla linea di velocità Salerno-Reggio Calabria, che rappresenta una connessione strategica per il Mezzogiorno. Insomma, siamo in presenza di una serie di interventi, di cui ho evidenziato solo i principali, per perfezionare la macchina amministrativa e dare un contributo alla crescita infrastrutturale così importante per lo sviluppo economico del nostro Paese. Trovo dunque strano che, all'inizio di questa seduta, ci si sia lamentati delle infrastrutture carenti nel nostro Paese, dei ritardi che ci sono nel nostro Paese, ma poi non si ammette che questo è un provvedimento utile per velocizzare il suo ammodernamento infrastrutturale, portarlo ancora più avanti e inserirlo degnamente in Europa. Per questi motivi

E lo fate evitando il dibattito. Lo fate, quindi, sapendo che potreste discutere di qualsiasi cosa qui dentro, perché avete i numeri per portare avanti qualsiasi cosa. Invece, la vostra continua ricerca di fiducia fa pensare che sia scatenata dal fatto che è proprio di voi stessi che non avete fiducia. Sottosegretario, del tempo che ci avete lasciato in Commissione per esaminare il decreto-legge: ben tre giorni. Io la ringrazio, davvero. Ovviamente sono sarcastica. Anche questo aspetto è figlio della vostra patologica e bulimica voglia di decretare, tanto che vi siete ritrovati a dover gestire un vero e proprio ingorgo prima della pausa Lasciatemi dire che tra una distrazione estiva e una olimpica, dove vi siete improvvisati anche esperti genetisti da bar dello sport e detentori di verità assoluta, una medaglia ve la siete meritata anche voi. Siete infatti riusciti a portare a casa la medaglia d'oro del vittimismo, che ormai avete eletto a sport nazionale. Come vittime, tra l'altro, vi siete presentati in occasione del quarantaquattresimo anniversario della strage neofascista di Bologna lo scorso 2 agosto, una strage per per cui sappiamo la verità e ne abbiamo le prove: furono la P2, i servizi segreti deviati e i neofascisti a ideare e a mettere in atto quel terribile attacco allo Stato, frutto di un preciso piano eversivo. Medaglia d'oro, quindi, al vostro vittimismo, ma la vostra faccia resta di bronzo per l'atteggiamento che mostrate di fronte alle verità che le sentenze e la storia ci consegnano proprio su questi fatti. Andiamo al merito del provvedimento: lo avete chiamato decreto infrastrutture, ma nel pentolone che è il testo di questo decreto-legge avete inserito tante di quelle materie che avreste fatto meglio a chiamarlo per quello che realmente è, ovvero un decreto *omnibus*. *omnibus*. Sì, perché si va dalla revisione del periodo regolatorio delle concessioni in scadenza, passando per le misure in materia di sport, fondazioni lirico-sinfoniche, scuole politecniche e modifiche al codice di procedura penale. Richiamate poi in questo decreto il Piano Mattei per l'Africa, grazie al quale distraete le risorse del Fondo italiano per il clima, per fare cosa ancora non è chiaro, perché non lo avete detto. Parliamo di un Fondo, quello italiano per il clima, nato per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici nel nostro Paese. In pratica avete deciso di utilizzare questo Fondo anche per investimenti nell'*oil and gas* che - come sappiamo tutti - sono tra le principali fonti di inquinamento atmosferico. E così, mentre aspettiamo che vi chiariate le idee su cosa fare per l'Africa lasciatemi dire che è all'Italia che servirebbe un Piano Mattei, sì, ma per le infrastrutture idriche, per renderci resilienti alla siccità, per eliminare gli sprechi, per far tornare l'acqua nelle case dei cittadini residenti in centinaia di Comuni italiani, per evitare agli agricoltori di mandare in fumo il loro raccolto. A me dispiace che oggi non sia qui presente il Ministro, perché volevo fargli i miei complimenti per suo tramite, Presidente, perché ricordo che all'incirca un anno fa lui varò il decreto siccità. Bene, complimenti: siamo ancora qui a parlare di questi problemi che quel decreto-legge non ha risolto minimamente. *(Applausi)*. Ad un certo punto, nella lettura di questo testo, troviamo un tema infrastrutturale, il vero tema dei temi che non poteva mancare: il Ponte sullo Stretto, certamente l'infrastruttura che risolve i problemi di tutti gli italiani al giorno d'oggi. È certo: è il chiodo fisso del ministro Salvini. E quindi leggiamo di importanti novità per i cittadini che ormai da un secolo sentono parlare di questa imponente e impattante opera.

proprio quello che ha riesumato il vecchio progetto per il Ponte; lo stesso progetto che è ancora in attesa della VIA e della VAS; lo stesso progetto che ancora attende di essere aggiornato con le 239 integrazioni richieste dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dicevo quindi di questa novità: la novità è che non approverete mai un progetto definitivo e lo scrivete nel testo del disegno di legge, perché prevedete che al suo posto vi saranno approvazioni per fasi costruttive, cioè a pezzetti, come se i lotti di un ponte non fossero tra loro funzionalmente dipendenti. Presidente, ma di cosa stiamo parlando? Voi state dicendo al Paese che procederete alla costruzione del Ponte sullo Stretto per lotti. Dite anche potrete terminare i lavori del lotto 2 senza che i lavori del lotto 1 siano terminati, perché appunto non dipendenti a livello funzionale. Mi domando però come si arrivi al lotto 2 se non passando dal 1. Attenzione: non sono io che sto dando i numeri. No: i numeri li ha dati e ben chiari il ministro Salvini, come se fosse ad una tombolata dell'ultimo dell'anno. Ad ottobre 2022 parlava di generazione di 120.000 posti di lavoro; poi nelle sue stime è iniziato a scendere, passando a 100.000

Infatti un'unità di lavoro annuo rappresenta la quantità di lavoro svolta da una sola persona impiegata a tempo pieno per un intero anno. Il Ponte non si realizza in un solo anno, ma ce ne vorranno almeno otto, almeno a detta del ministro Salvini. Voglio però aggiungere un altro anno, perché non si sa mai se vi saranno i ritardi che sono scritti in questo decreto-legge sono già dichiarati. Aggiungiamo comunque un altro anno e diciamo che il Ponte si realizzerà in nove anni. Allora, Ministro, sarebbe stato molto più semplice prendere quel dato, cioè le 120.000 unità di lavoro annue, e dividerlo per nove, che sono gli anni previsti per la realizzazione del Ponte. Avrebbe ottenuto così la stima dei posti di lavoro attivabili. È una semplice questione matematica, quella scienza esatta lontana anni luce dal ministro Salvini. Un Ministro, Presidente, che è sparito dai *radar* e che nulla dice dei veri problemi che in questi giorni stanno facendo agonizzare il sistema dei trasporti italiano, da quello ferroviario a quello aeroportuale. Quello che mi chiedo e che avrei avuto piacere di chiedere al ministro Salvini è che cosa ne pensa dell'impatto che i cantieri sulla linea ferroviaria stanno generando e continueranno a generare sul servizio. Che cosa ci direbbe lui su quello che è accaduto nelle ultime settimane, ovvero dei pesanti disagi e delle interruzioni che hanno compromesso per ore, se non per giorni, diversi tratti della rete dorsale? Parlo dell'incidente ferroviario del 9 luglio sulla linea Salerno-Paola, di quello dell'11 luglio a Parma, sulla linea Milano-Bologna, dell'inconveniente del treno merci adibito al trasporto auto, che in data 18 luglio ha perso le auto che trasportava lungo la linea dei binari, e e delle numerose anomalie e dei guasti che hanno messo duramente in crisi tutte le dorsali principali. accettato a buon cuore la richiesta dei colleghi delle opposizioni di chiedere al ministro Salvini di venire a riferire su questi fatti, come abbiamo fatto anche la settimana scorsa affidandoci a delle note stampa. però un altro punto, un altro dato che è stato reso noto da poco dall'osservatorio ASAPS, che riguarda la sicurezza stradale, e anche su questo sarebbe utile che il Ministro si aprisse ai cittadini. Dal punto di vista della sicurezza stradale, luglio è un mese tragico per le morti, avendo contato un morto al giorno sulle strade. I decessi dall'inizio dell'anno sono 232. Parliamo di persone uccise anche nel momento in cui stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. addirittura di persone che camminavano sui marciapiedi. Avrei chiesto al Ministro, se fosse stato presente oggi, al netto di quello appena detto, se ritiene ancora opportuno continuare a concentrare la sua attenzione e quella dei suoi uffici sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. In conclusione, Presidente, mi rivolgo al

la vostra fortuna politica, alimentandola poi con ridicolo vittimismo e prevedibile narcisismo. Voi volete dividere e spaccare, perché è l'unica cosa che vi riesce di fare, ma il Paese non ha certo bisogno di questo. Per questo e tanti altri motivi, Presidente, annuncio il voto contrario del mio Gruppo sulla questione

non farò una difesa d'ufficio del ministro Salvini, perché non ne ha bisogno e anche perché mi rendo conto che le opposizioni devono fare il loro mestiere, visto che non hanno argomenti o non riescono a incidere sui provvedimenti. Quindi, a differenza di chi vorrebbe chiudere il Parlamento per per andare a fare il bagno al mare, siamo orgogliosamente - io, il Gruppo della Lega e tutta la maggioranza - qui il 5 agosto per la conversione di un decreto-legge che riteniamo importante per l'Italia e per lo sviluppo per lo sviluppo delle infrastrutture. Si tratta di un decreto-legge con pochi articoli, però importantissimo per tante opere strategiche del Paese, perché sblocchiamo opere indispensabili e attese da anni che rischiavano di rimanere incompiute nel tempo a causa del caro prezzi o - come spesso accade - per la complessità dell'*iter* burocratico. È un decreto-legge che spazia da disposizioni in materia di concessioni autostradali al Ponte sullo Stretto - come più volte richiamato in quest'Aula - ancora una volta però per perfezionare l'*iter*, proprio visto l'imminente avvio dei cantieri. Vi è poi un articolo che prevede anche un piano di razionalizzazione sui commissari straordinari degli interventi infrastrutturali. I commissari non sono un capriccio, ma servono ad accelerare le infrastrutture e le opere ritenute prioritarie. È prevista la revoca dei commissari che già hanno finito il loro compito, e hanno terminato hanno terminato la realizzazione dei cantieri, e la nomina di nuovi commissari in base anche alle nuove esigenze. Nei vari articoli possiamo trovare moltissime opere che saranno finanziate e sburocratizzate, e interventi che vanno da Nord a Sud

piuttosto che ai 150 milioni di euro per il sistema idrico del Peschiera. In un momento in cui - ve lo dico da siciliano - stiamo vivendo un dramma in Sicilia per la siccità in una terra dove da più di un anno non piove, mi pare sia urgente e importante parlare di un sistema idrico che porterà l'acqua all'acquedotto di Roma. Penso ai quasi 400 milioni di euro per il collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, e di conseguenza - chi ha visione fa anche questo alla proroga dei termini per l'adozione dei decreti di esproprio per il completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e, quindi, del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, tanto caro al nostro sottosegretario Durigon. Penso a quanto contenuto in questo decreto-legge sull'opera ingegneristica più importante del secolo: non è uno dei tanti cantieri, ma sarà il più importante che questo Governo, il nostro Paese e il mondo intero avranno da osservare. Grazie all'entrata in vigore di questo decreto-legge finalmente si potrà approvare il progetto esecutivo e si potrà approvare per fasi costruttive,

che accerterà l'esistenza della copertura per l'intero fabbisogno dell'opera. Ovviamente la copertura c'è, ma verrà accertata nel momento in cui il progetto verrà approvato. È una progettazione esecutiva che ha l'obiettivo di ottimizzare la costruzione della struttura contenendo tempi e costi. La fattibilità tecnica dell'opera non è mai stata messa in discussione o è stato fatto soltanto magari dai soliti detrattori dopo anni di chiacchiere e di attese, grazie finalmente a questo Governo e all'impulso che ha voluto dare il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, si sta finalmente concretizzando la realizzazione di questa straordinaria opera, che non è importante soltanto per Messina o per Reggio Calabria, ma è importante per l'Italia intera e strategica per l'Europa, per l'intero Mezzogiorno, per la Sicilia e per la Calabria. In più, vi sono 40 milioni di euro, sempre legati al Ponte sullo Stretto, stanziati per gli espropri delle abitazioni che sono ubicate dove verranno realizzati i cantieri, ossia nella zona di costruzione; milioni di euro che giustamente serviranno per i cosiddetti espropri bonari, con cui per legge si prevede anche una maggiorazione del 15 per cento del valore immobiliare. Come è giusto che sia, per il caso di esproprio di un immobile adibita ad abitazione principale, al proprietario viene riconosciuta una indennità aggiuntiva. Strumentalmente e vergognosamente assistiamo a uno sciacallaggio delle sinistre e delle opposizioni che fanno soltanto demagogia, perché non hanno altro da fare in questo momento, dicendo che il Ponte adesso non si potrà realizzare perché c'è la siccità.

il ministro Salvini, facendo una ricognizione dei progetti presentati, ha finanziato un miliardo dei fondi in dotazione del MIT, di cui ben il 10 per cento specificatamente in opere per la Sicilia. vorrei ricordare un altro emendamento approvato alla Camera dei deputati, a prima firma dell'onorevole collega Anastasio Carrà, vice presidente della Lega in Sicilia: un emendamento che siamo riusciti a inserire all'articolo 3,

del porto di Tremestieri, un cantiere chiuso da anni. Grazie a questo Governo, grazie a questo Ministro e grazie ai Sottosegretari, viene finanziata la piattaforma logistica del porto di Tremestieri, strategica perché, in attesa dell'attraversamento stabile dello Stretto,

chiudendo una stagione fallimentare dei no che ha causato una notevole carenza di infrastrutture nel nostro Paese. Questa è la Lega. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier.

ferrovie in panne, linee sotto stress, avarie e guasti, come il blocco di 350 persone a Grosseto senza aria condizionata e i 300 passeggeri bloccati a Napoli; sulla linea ad Alta Velocità Roma-Firenze vi sono stati undici episodi di problemi tecnici in soli dieci giorni centinaia di voli saltati per avarie tecniche. La settimana dal 15 al 21 luglio ha visto la puntualità dei voli crollare al 49,7 per cento, con l'Italia che rappresenta il 15 per cento di tutti i ritardi europei. Più volte è stato chiuso l'aeroporto di Catania, causando cancellazioni e ritardi. Anche la cerimonia inaugurale alle Olimpiadi a Parigi ha visto oltre 2.500 passeggeri italiani bloccati, con risarcimenti stimati in 1 milione di euro. Per non parlare delle code interminabili in autostrade e delle mega file nei porti; la Calabria bloccata per cinque giorni; lunghe code a Pavia, treni bloccati per oltre sei ore ; code, blocchi e ritardi sono all'ordine del giorno sulle autostrade liguri ormai da diversi anni. La linea Alta Velocità Milano-Bologna sarà parzialmente interrotta dal 12 al 18 agosto, con un aumento dei tempi di percorrenza fino a due ore. Il caos trasporti in Italia durante l'esodo estivo è solo un segnale d'allarme. Serve un intervento urgente per garantire la mobilità dei cittadini e la competitività del nostro Paese. Come risponde a questa emergenza, al caos totale dei trasporti, il Governo? Con questo decreto, un decreto-legge minestrone senza una visione, senza programmazione né pianificazione delle opere. Vi sono risposte a questi problemi? Vi sono almeno le basi per affrontare il problema e superarlo? No, nulla di tutto ciò. Certo, vi sono alcune misure spot utili e, quando si fa qualcosa di giusto ed importante, avrete sempre il nostro sostegno, perché siamo all'opposizione, ma siamo un'opposizione che agisce nell'interesse del Paese. Leggendo l'elenco di interventi, ve ne sono certo alcuni che, presi singolarmente, ci trovano d'accordo, come il parziale finanziamento del trasporto pubblico locale, la bonifica del sito di interesse nazionale a Cogoleto-Stoppani, o il finanziamento del Parco scientifico tecnologico di Erzelli. Ma, se il tema era finanziare in maniera indistinta le opere presenti nel territorio, che hanno bisogno di interventi urgenti, perché non avete accolto le molte proposte del Partito Democratico presentate in Commissione alla Camera e al Senato? Parlo delle nostre proposte per sostenere il trasporto pubblico di tutta l'Italia per sopperire alle carenze infrastrutturali, come ad esempio la Tirrenica per il Lazio e la Toscana, in particolare per quei lotti già cantierabili ; per il rafforzamento dell'Autorità di bacino del Po, dove chiedevamo personale aggiuntivo per poter portare avanti i progetti ; per l'interporto di Termini Imerese ; i ponti sul fiume Po, il ponte di Parma, il ponte sul torrente Stura a Campo Ligure ; il ripristino del finanziamento dei fondi tagliati alla tramvia di Firenze ; il finanziamento del Fondo nazionale del trasporto pubblico, così come del Fondo per il contratto nazionale degli autoferrotranvieri ; le risorse aggiuntive per le metropolitane di Roma Capitale ; i maggiori finanziamenti per il trasporto aereo della Sicilia ; nuove risorse per i collegamenti insulari, in in particolare per mantenere la continuità territoriale in certe isole, soprattutto quelle più piccole. Come vedete - lo dico ai colleghi di maggioranza che sono intervenuti - abbiamo fatto tante, numerose, diverse proposte. E ancora - lo dico per la terra da cui provengo - la richiesta, ormai riproposta da due anni, dell'esonero del pedaggio per i transiti delle autostrade liguri, considerando i disservizi dovuti ai cantieri interminabili. In teoria è una proposta condivisa da tutte le forze politiche, quando parlate sul territorio, ma sempre bocciata qui a Roma, quando si tratta di passare dalla propaganda ai fatti. dico nessuno di questi emendamenti è stato approvato. Perché non erano necessari e urgenti? No: perché avete destinato tutte le risorse a un progetto, quello del Ponte, che aspetta ancora la risposta a oltre 200 prescrizioni, ma che per voi è propaganda e vale più delle emergenze reali. Ne ha già parlato bene in dettaglio il collega Fina: non solo il costo di quest'opera preclude il finanziamento a centinaia di interventi urgenti in tutta Italia, soprattutto al Sud Italia, ma la scelta fatta in questo decreto delle fasi costruttive rischia di dare un'ulteriore svolta in negativo. Potreste essere il primo Governo di destra che, oltre a sprecare un sacco di soldi per parlare del Ponte sullo Stretto, sprecherà altri soldi pubblici per lasciare ecomostri destinati per secoli a ricordarci quanto sia stata sventurata la scelta di avventurarsi in un'impresa senza la dovuta serietà. I cittadini calabresi e siciliani davvero non se lo meritano. Peccato: poteva essere l'occasione per dare una risposta di sistema, per affrontare un'emergenza vera che gli italiani stanno vivendo ogni giorno. Noi non abbiamo fatto quello che faceva il ministro Salvini quando era all'opposizione. Non siamo andati nelle stazioni a fare i video, a strumentalizzare i cittadini che stavano lì, cercando di trovare il modo di vivere quei pochi giorni di vacanza che avevano ritagliato proprio in queste settimane e che, invece di passarli nelle località di villeggiatura, li hanno dovuti passare nelle stazioni, aspettando servizi sostitutivi di cui non erano stati informati, con temperature incandescenti. Non siamo andati a raccogliere il disagio per alimentare bestie e bestioline *social*, per alimentare disagio. Noi non abbiamo fatto questo. Noi abbiamo chiesto al ministro Salvini di venire a riferire in Parlamento, di venirci a spiegare cosa sta facendo e cosa non sta facendo. Noi pensiamo che, se va per aria il sistema dei trasporti del Paese, non è un problema solo di questo Governo, ma è un problema di tutte le istituzioni, è un problema del Parlamento. Voteremo no alla fiducia, perché il Governo e il Ministro non possono continuare a scappare dalla realtà e occuparsi solo di dibattiti ideologici o di richiami revanscisti a epoche buie del nostro Paese. Stia tranquillo il ministro Salvini, che anche oggi non è presente: per lui non varrà neppure il falso storico. Di lui nessuno dirà mai, in futuro, che, quando c'era lui, i treni arrivavano in orario.

avevo fatto una promessa: mi ero imposta - forzatamente, con il mio carattere - di non commentare più le sventure dei Governi che ci hanno preceduto; di non parlare del decennio *horribilis* in cui, pur di rimanere attaccati alle poltrone, le attuali forze di opposizione - sempre per fortuna opposizione - senza una visione senza un progetto di Nazione, senza un minimo, avrebbero stretto accordi anche con Attila per rimanere lì. Ma purtroppo i cantori di questa sinistra, che con la solita, metodica insolenza discettano sui problemi del mondo sempre da qualche spiaggia di Capalbio o al fresco di qualche valle che licenziano verdetti e non decreti, con tanta ironia nei nostri confronti, mi costringono a rompere il giuramento. Mi costringono a riprendere il filo di un discorso logico che pare loro sfuggire, consapevolmente o meno e forse nemmeno tanto in buona fede. fede. Dalle pagine del «Corriere della sera», uno dei capocomici della compagnia dei cantori, tra un caffè annoiato e un bicchiere di *champagne* svampito, ha stigmatizzato l'operato di un dirigente dell'Alta velocità, reo, secondo la sua tesi, di aver programmato lavori sulla rete nel periodo estivo, penalizzando il traffico e la stagione turistica. Si tratta di un'altra serie di strafalcioni in cui spiccano grossolane imprecisioni, tipiche di chi parla senza cognizione di causa, con il solo intento di screditare (per il piacere di ricevere dei *like* di qualche profilo *fake* creato appositamente) chi, invece, lavora concretamente per il bene della nostra Italia. Non sapere e forse volutamente ignorare che le interruzioni per lavori non sono decise dalle imprese ferroviarie (nel caso specifico dell'Alta velocità) è veramente grave. I lavori di manutenzione straordinaria e quelli per la realizzazione di grandi opere sono programmati e gestiti dal gestore dell'infrastruttura Rete ferroviaria italiana. Con rammarico anche questa volta ci rendiamo conto che la conoscenza del sistema Italia non è nelle corde di chi vive nella bolla delle zone completamente sconnesso dai problemi del vivere quotidiano e del mondo; quel mondo reale che viene affrontato concretamente dal Governo Meloni attraverso questo decreto-legge, che, ad esempio, all'articolo 3 specifica i criteri relativi alle nomine dei commissari, tenendo conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti. Anche su questo dovevamo arrivare noi. Mettiamo un punto, però, e affrontiamo la situazione reale. Solo per fare qualche esempio, in questa cornice saranno realizzati il nodo di Genova e il terzo valico dei Giovi; la linea Alta velocità-Alta capacità sulla tratta Milano-Verona; la tratta Brescia-Verona-Padova, che comporterà una velocizzazione dei treni e la costruzione di stazioni ad esclusivo utilizzo dell'Alta velocità a Verona e Vicenza; la linea Alta velocità-Alta capacità sulla tratta Napoli-Bari; il raddoppio in variante di circa 20 chilometri di linea della tratta Apice-Hirpinia; il raddoppio in variante della tratta Hirpinia-Orsara-Bovino, con la nuova stazione di Hirpinia; il potenziamento della linea Venezia-Trieste nel tracciato Venezia Mestre-Ronchi Sud. Solo chi, come me, proviene da quelle zone conosce i benefici di un'opera al centro dell'Europa, che stiamo attendendo da tempi immemori. il passante Alta velocità-Alta capacità di Firenze e la nuova stazione di Belfiore, dotata di *hub* intermodale, in connessione con la stazione di Firenze Santa Maria Novella, tramite *people mover* dedicato, e con l'aeroporto di Firenze tramite la linea tranviaria; il potenziamento della linea adriatica che permette, insieme alle opere elencate, di collegare le Regioni adriatiche con il centro dell'Europa; la la realizzazione della nuova tratta Battipaglia-Romagnano, con benefici immediati per i collegamenti su Potenza, e la tratta Romagnano-Praia, con una confluenza dell'attuale linea tirrenica (parliamo dei famosi collegamenti). Sia chiaro, non mi è stato alcun segreto di Stato; ho avuto solo la curiosità - che è mancata a certi colleghi che mi hanno preceduto e ai giornalisti di certa stampa - di informarmi, banalmente (non sono un genio) sui siti istituzionali, ma quest'attività e soprattutto la conoscenza dello stato dell'arte avrebbe compromesso la possibilità, per la stampa al soldo dell'opposizione, di dispensare le critiche sull'attività del Governo e non avrebbe soddisfatto la parte politica che sostengono e che li sostiene. Avrebbe impedito loro di mistificare la narrativa e di cavalcare la propaganda disfattista. Questa volta, però, nel cavalcare la propaganda si è precipitati nel ridicolo, non solo confondendo grossolanamente ruoli e funzioni, ma colpendo ingiustamente e colpevolmente chi giornalmente è impiegato con professionalità a far funzionare una parte fondamentale della mobilità. È evidente una volta in più, riprendendo il pezzo da cui ho tratto spunto, come vi sia una parte, per fortuna ristretta, di soggetti che sono del tutto estranei al quotidiano, al mondo del lavoro e ai problemi della gente. Determinati lavori, come quelli di cui vi state lamentando e che vi ho letto, vanno fatti nel periodo in cui l'attività lavorativa generalmente indicata - fabbriche, scuole o attività produttive - è sospesa, per creare il minor disagio al sistema Paese, un po' come succede in tutte le parti del mondo. Un mondo che non è circoscritto nei salotti e nei circoli, perché anche dei problemi dei teatri e dei lavoratori dei teatri ci stiamo occupando noi in questo decreto. Un mondo reale ha un raggio d'azione molto vasto (lo ridico, banalmente, sempre per lo stesso motivo di prima): mi riferisco alle attività produttive, alle scuole o alle fabbriche; ciò non significa mortificare e penalizzare una parte importante del nostro PIL, il turismo, ma bisogna avere coraggio, quello che vi è mancato negli ultimi dieci anni, perché questo significa governare, ossia avere coraggio di fare delle scelte, guardando al futuro della Nazione e non alla gestione spicciola, che, come si è visto, penalizza tutti, in particolare l'Italia. Sarebbe onesto, ma mi rendo conto che questa parola non appartenga al vocabolario di certa sinistra e della sua stampa, che prima del prossimo caffè partisse una lettera di scuse a quegli uomini e a quelle donne, a quei dirigenti e a quei lavoratori che in questo difficile periodo sono in prima linea per assicurare che alla ripresa *post*-ferie - sempre le ferie degli altri, a Capalbio - scuole, fabbriche, attività e anche i teatri, appunto, possano riprendere senza troppi disagi. *(Applausi)*. Sono conscia che né la vergogna, né la consapevolezza dei propri errori, come i banchi a rotelle mi suggeriscono *(Applausi. Commenti)*, appartengano al DNA di soggetti che per lunghi anni, quantomeno appunto i dieci di cui sopra, non hanno visto l'elefante nella stanza. Lo dico senza polemiche: tornate o rimanete nel vostro riposo onirico, noi continueremo responsabilmente a lavorare per la gente, con la gente. Pertanto, esprimo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Avanti così.

con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

*(Commenti).* Come ho già preannunciato, non ci possono essere in questo momento gli interventi di fine seduta, perché la seduta non è terminata, ma è sospesa in attesa degli esiti della Conferenza

Signora Presidente, in queste settimane ricorre il centenario della nascita di Danilo Dolci, definito in vario modo sociologo, poeta, educatore, attivista attivista politico della non violenza. Fu soprannominato anche il Gandhi italiano. Molti di noi lo ricordano soprattutto per le grandi battaglie che fece in Sicilia: partendo dal Nord, dopo aver disertato negli anni del fascismo ed essere stato arrestato dai nazifascisti, scelse la Sicilia, tra Trappeto e Partinico, come luogo nel quale avviare alcune delle esperienze che aveva maturato nel Nord Italia, in particolare creare delle comunità dedicate ai bambini e ai bisogni degli ultimi. Creò un borgo, il cosiddetto Borgo di Dio, dedicato appunto ai bambini, e iniziò un'attività di educazione molto particolare nella quale inventò l'autoanalisi popolare, cioè l'idea di

C'è una frase molto bella di una sua poesia che recita: «C'è chi educa sognando gli altri come ora non sono, ciascuno cresce solo se sognato». un'iniziativa, un'attività che ebbe grande risalto in tutta l'Italia. Per esempio, il 14 ottobre 1952 iniziò uno sciopero della fame sul letto di Benedetto Barretta, un bambino morto per la denutrizione. Nel 1956 avviò uno sciopero della fame collettivo contro la pesca di frodo e le autorità del tempo giudicarono quel digiuno pubblico come illegale. Poi iniziò nel 1956 lo sciopero alla rovescia: sciopero alla rovescia: di fronte alla carenza di infrastrutture in cui versava in quel momento la Sicilia, lui decise di avviare assieme ad altri disoccupati un'attività per costruire una strada laddove non c'era. Danilo Dolci fu arrestato. Si ebbe un processo che attirò tantissime persone, tra le quali Carlo Levi, Elio Vittorini e tanti altri che testimoniarono quell'attività. Fu difeso da Calamandrei, che parlò di lui come l'uomo di cultura l'uomo di cultura che, per manifestare la sua solidarietà ai poveri, non si è accontentato della parola parlata o scritta, dei comizi, degli ordini del giorno e dei messaggi, ma ha voluto vivere la loro vita, soffrire la loro fame, dividere il loro giaciglio, scendere con loro nella forzata abiezione per aiutarli. Ricordiamo anche in questi giorni la grande protesta che fece per l'acqua in Sicilia, fino alla costruzione della diga dello Jato. A quel proposito, quel proposito, Danilo Dolci a proposito dell'acqua disse che «l'acqua può divenire non soltanto occasione per elevare la produttività e il reddito, ma anche leva di cambiamento strutturale per un cambiamento della struttura di La lotta per l'acqua, la lotta per l'uguaglianza, la lotta per i diritti dei più poveri: questioni assolutamente attuali che ci fanno pensare a Danilo Dolci non soltanto come un testimone, ma come qualcuno che ci sta suggerendo ancora una lezione per liberare dai bisogni le nostre popolazioni. Grazie, senatore Nicita, per aver ricordato un processo storico a cui diede inizio, perché quell'arresto fu dovuto al fatto che erano in vigore i testi unici di sicurezza del ventennio fascista precedente. Da quel processo in poi inizia una lettura costituzionalmente orientata delle norme ancora in vigore

una collega mi chiede di fare questo intervento in Aula per lei. Una richiesta così non capita spesso, ma è importante, perché significa: mi fido di te, so che interpreterai il mio pensiero. È per questo che ho detto subito di sì alla collega Antonella Zedda e quindi questo è il mio intervento, ma è anche il suo. Le donne sono forti quando sono unite. Anche questo non capita spesso, ma, quando si riesce a fare squadra, i risultati sono notevoli, come nel caso di Francesca Deidda. La storia è nota a tutti. Questa ragazza di San Sperate, in provincia di Cagliari, viene uccisa in casa con un colpo alla fronte; poi il corpo viene messo in un borsone e abbandonato in campagna. Il marito si professa innocente e, all'inizio, non vi sono elementi a suo carico. C'è però la *chat* che Francesca aveva con le colleghe del *call center* per il quale lavorava. Le colleghe rilevano subito alcune anomalie dopo le dimissioni dal lavoro della donna e la contattano per chiederle i motivi della decisione. Ma le risposte arrivano soltanto via WhatsApp e il tono dei messaggi accresce i dubbi. Non può essere lei che scrive «voglio stare da sola, non voglio vedere nessuno, mi isolerò per un po' di tempo». E allora mettono in atto una strategia, per scoprire se chi scrive sia proprio lei. Inventano il nome di una collega, scrivendo che si è dimessa anche lei; e la risposta che arriva è: «mi dispiace, come mai?». L'autore del messaggio è caduto nella trappola; è chiaro che non può essere Francesca, che avrebbe certamente saputo che il nome di quella collega era inventato. Da qui iniziano le indagini ufficiali, che si dirigono verso il marito, che viene arrestato. Le donne che si uniscono e fanno rete. Non capita spesso, è vero; ma, quando accade, i risultati sono straordinari. Forse è questa la chiave per reagire alla violenza: attivarsi per un'amica, mettersi nei suoi panni, fare ciò che siamo certe lei farebbe per noi. Empatia, solidarietà, è questo che ci rende forti. E allora impariamo a fare rete, a restare unite, a restare forti. Grazie, senatrice Campione. Le parole su questi episodi non sono mai abbastanza.

La seduta di domani prevede la discussione del decreto-legge in merito alle materie prime critiche di interesse strategico e dei disegni di legge Rendiconto 2023 e Assestamento 2024, Grazie, i lavori delle Commissioni riprenderanno a partire da martedì 3 settembre, ferma restando la possibilità di convocarsi anche in precedenza in relazione a situazioni di urgenza connesse con le materie di propria competenza. L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 11 settembre, alle ore 16,30, per la discussione di ratifiche di accordi internazionali. Si è stabilito che l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della Rai avverrà alla ripresa dei lavori dell'Assemblea, ragionevolmente il giorno 12, previ accordi con la Camera dei deputati. Il calendario della settimana prevede inoltre, giovedì 12 settembre, il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*. Il calendario dei lavori potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e concernenti semplificazione e digitalizzazione di attività economiche e servizi, nonché semplificazione normativa e qualità della normazione.